"Il link apre una nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Onorevoli colleghi, vi informo che non è ancora pervenuto il parere della 5a Commissione permanente sul disegno di legge concernente il riconoscimento della lingua italiana dei segni.

mi rivolgo a lei, ai colleghi senatori e alla Sottosegretaria presente. Il disegno di legge che stiamo esaminando, che è stato presentato in Commissione qualche tempo fa, non è particolarmente complesso e anche la relazione sarà quindi assolutamente breve.

di un tema molto sentito, soprattutto nell'ultimo periodo, tanto a livello internazionale quanto a livello nazionale e cioè la lotta alla corruzione. Non mi soffermo, perché ne abbiamo parlato molte volte in quest'Aula e in Commissione, su quanto il fenomeno della corruzione abbia preso piede, però voglio sottolineare che, in modo altrettanto fermo e deciso, il nostro Parlamento ha adottato una serie di provvedimenti estremamente incisivi e duri per contrastare tale fenomeno. Abbiamo trattato della Abbiamo trattato della corruzione in numerosi altri settori, in particolare nel settore della pubblica amministrazione, abbiamo approvato alcuni provvedimenti che sono già entrati a regime e che stanno producendo sicuramente effetti importanti.

si tratta di persone che svolgono un'attività giurisdizionale o comunque attività giudiziarie in genere, dato che in Commissione abbiamo ampliato la platea delle persone che possono rispondere di questi reati,

all'ordinario comportamento, che pure richiede la medesima onestà, liceità e affidabilità. Ripeto che, da una certa categoria di persone, ci si aspetta un atteggiamento sicuramente molto più concretamente affidabile rispetto ad altre categorie. Questo è il tema che viene affrontato dal disegno di legge

L'articolo 1 introduce un'aggravante all'articolo 317 del codice penale, relativamente al reato di concussione. In base alla norma, per il reato di concussione è previsto un aumento della pena fino alla metà, qualora i fatti corruttivi siano stati commessi in relazione all'esercizio di «attività

e cioè l'induzione indebita a dare o promettere utilità, nel caso in cui tali reati vengano commessi, ancora una volta, in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

il soggetto attivo appartenesse alla platea delle persone che ho richiamato in precedenza. L'ex articolo 3, oggi 4 a seguito dell'introduzione del nuovo articolo 3, reca una nuova circostanza aggravante per il reato di millantato credito. caso le pene sono aumentate fino alla metà se i fatti previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Come noto, l'articolo 346 del codice penale prevede due distinte ipotesi delittuose, con differente struttura e configurazione, rispettivamente nei commi primo e secondo. La fattispecie di cui al primo comma, sanzionata con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a 2.065, consiste - per specificarlo meglio - nel millantare credito per farsi

consiste nel farsi retribuire con il pretesto di dover comprare il favore di un pubblico funzionario o di doverlo remunerare. Anche in questo caso la pena, quando compiuta dai soggetti che ho più volte richiamato, viene aumentata fino alla metà. articolo 4, oggi articolo 5, ultimo di questo disegno di legge, interviene invece sul reato di traffico di influenze illecite. Si tratta di un tema che nell'ultimo periodo è stato oggetto di importanti discussioni; un tema

di prevedere lo stesso aggravamento di pena, e cioè l'aumento fino alla metà, qualora le condotte illecite vengano poste in essere, ancora una volta, dai soggetti

il provvedimento in titolo sia di estrema importanza. È per questo che nel corso dei lavori in Commissione si è deciso di rivolgere particolare attenzione al tema e si è lavorato molto anche per cercare di renderlo il più omogeneo possibile rispetto al sistema. Credo che questo lavoro sia riuscito anche bene e di questo bisogna ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, maggioranza e opposizione, in maniera molto fattiva

con noi parlamentari.

di un provvedimento che introduce aggravanti di pena - come ha detto con molta onestà intellettuale il relatore - per i reati commessi in riferimento ad attività giudiziarie. Questo ci deve innanzitutto interrogare, perché qui, prima di votare i provvedimenti,

In primo luogo, esso nasce in una fase storica in cui sicuramente si sono registrate molte vicende giudiziarie che hanno riguardato magistrati, avvocati e operatori della giustizia in senso lato e quindi non colma affatto

non si affida al magistrato, che può sempre, tra un minimo e un massimo della pena, valorizzare ai fini della quantificazione della sanzione le qualità soggettive, la particolare competenza e la particolare responsabilità

ci sarà stato un filo conduttore che ha portato la Commissione alla qualificazione di questi reati anziché di altri, ci sarà stato un motivo per questa selezione. Certamente si tratta dei reati in cui più facilmente può incorrere un operatore della giustizia e questo sarà il motivo per cui sono stati elencati

introduce modifiche agli articoli 317, 319-*ter*, 319-*quater*, 346 e 346-*bis* del codice penale. Stiamo parlando dei reati di concussione, di corruzione in atti giudiziari, di millantato credito e di traffico di influenze illecite. In sostanza, il provvedimento introduce aggravanti di pena per i casi in cui la commissione dei reati avvenga da parte di coloro che svolgono la professione forense ovvero esercitano attività giurisdizionale cosiddetta di prossimità

parla in maniera molto chiara e condivisibile di lotta alla corruzione. Nella relazione si dice in modo lineare che la corruzione rischia di divenire un un fenomeno ambientale ed endemico e «di determinare, nel tempo, una sorta di perversa abitudine alla corruttela». Questo è il rischio, se non si interviene con strumenti efficaci per contrastare i fenomeni corruttivi.

Avremmo potuto scriverla noi questa premessa, però non stiamo parlando di strumenti efficaci per contrastare la corruzione:

Si vuole contrastare il fenomeno della corruzione intervenendo con un provvedimento che non prende neppure in considerazione il cuore del problema. Noi abbiamo cercato di dare il nostro contributo per migliorare il provvedimento. Abbiamo depositato degli emendamenti. Li illustro brevemente, ma avremo occasione di approfondirli. Innanzitutto l'emendamento 1.1, che prevede una riforma dei termini di prescrizione, perché possiamo avere tutte le leggi per contrastare i fenomeni corruttivi che vogliamo,

Sospendendo il termine di prescrizione, avremmo innanzitutto la certezza della pena, tempi più rapidi e processi più brevi, perché si farebbe molto più ricorso

Cos'è il Daspo? È una pena accessoria che abbiamo proposto molte volte nelle Aule del Parlamento; essa prevede l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione per chi si è reso colpevole, con sentenza passata in giudicato, di reati gravi nei confronti della pubblica amministrazione.

infatti, ieri, alla Camera dei deputati, il Partito Democratico ha bocciato la proposta di istituzione con urgenza della Commissione di inchiesta sulle banche. E dico questo per ricordare la credibilità di certe dichiarazioni. Non c'è solo la prescrizione, non c'è solo il Daspo. Noi abbiamo proposto un emendamento a questo provvedimento che consenta le cosiddette operazioni sotto copertura. Spesso il Movimento 5 Stelle - e non é il solo - si è dichiarato a favore di questa importante innovazione, per fornire agli inquirenti degli strumenti efficaci per fare emergere il fatto corruttivo. E questo é uno strumento che funziona molto bene in molti Paesi e noi, che abbiamo un problema della corruzione maggiore, invece non lo utilizziamo. Perché? Ma vogliamo veramente contrastare i fenomeni corruttivi? Allora, se vogliamo veramente contrastare il fenomeno corruttivo, perché lasciamo prendere la polvere alla proposta di introdurre nel nostro Paese

Dobbiamo fare una riforma del falso in bilancio, che è un reato gravissimo. Si pensi ai danni che ha procurato. Io sono veneto e vengo da Vicenza, dove c'è la sede della Banca Popolare di Vicenza. A Treviso, invece, c'è Veneto Banca. Parliamo di falso in bilancio e parliamo di 200.000 famiglie ridotte sul lastrico. Possiamo parlare della riforma del 416-*ter*: no a qualsiasi alleanza tra mafia e politica. L'attuale formulazione è inefficace, e lo sappiamo. Allora riformiamolo. Vogliamo parlare di autoriciclaggio e della sua riforma che, di fatto, non affronta, se non in misura minima, il problema di questo reato nel nostro Paese? In conclusione, di cose da fare ce ne sarebbero moltissime per contrastare efficacemente il fenomeno della corruzione nel nostro Paese. Ma, ancora una volta, di tutto ciò che ho citato fino adesso non facciamo nulla. Allora, forse, questo provvedimento serve per mettere una bandierina e per poter dire che abbiamo fatto qualcosa, come se il problema della corruzione in Italia fosse riferibile agli avvocati e ai cancellieri. Con l'approvazione anche di uno solo degli emendamenti da noi proposti potremmo dare una significativa accelerata alla lotta alla corruzione nel nostro Paese.

una volta, la cosiddetta montagna che partorisce un topolino: un provvedimento magari anche condivisibile, ma inutile sul piano del contrasto alla corruzione nel nostro Paese.

perché questo provvedimento? La ragione è semplicissima: quando abbiamo trattato i reati di corruzione e concussione

non si è pensato di immaginare delle aggravanti quando i soggetti che si rendevano responsabili di tali reati appartenessero a una determinato categoria di operatori del nostro Paese.

no. Il provvedimento in esame non sottende affatto un sospetto verso la magistratura. Anzi, io credo che sia la certificazione

tutti vengono colpiti da un immaginario collettivo che vede corruzione e reati commessi a qualsiasi livello da qualsiasi organismo statale. Ebbene, nei confronti della magistratura è un'attività preventiva. Se crolla anche questo pilastro importante della democrazia di un Paese, allora davvero siamo allo sfascio. Immaginare, quindi, delle aggravanti per tutti coloro che, operatori del diritto, garantiscono e danno garanzia di democrazia, di equità e giustizia nel nostro Paese significa proprio questo.

Io credo che un magistrato che ha lavorato e operato per trenta o quarant'anni nell'ambito della giustizia e ha servito lo Stato in quel settore non possa, possa, nel momento in cui viene collocato in pensione, avere una considerazione diversa rispetto a quella che era la considerazione di se stesso quando faceva giustizia nel nostro Paese.

di garanzia per i cittadini e di maggiore autorevolezza della stessa magistratura. Per queste ragioni, il Gruppo

per qualcosa che forse non merita la nostra attenzione. Questa è una valutazione personale. Io credo che quello della corruzione, della concussione e dei reati contro la pubblica amministrazione sia un tema di attualità

Quindi, non comprendo per quale ragione possiamo fare leggi che contrastano la corruzione, trascurando di considerare una sorta di ossequio e rispetto per gli amministratori del nostro Paese, che pur meritano, e dovremmo invece bloccarci nel fare lo stesso nei confronti di una categoria di operatori del diritto. che non possa esservi opposizione a un provvedimento come quello in esame che salutiamo con favore e voteremo di qui a poco con convincimento.

un rilevante aggravio di pena, possa rivolgere, sia pure a due vecchietti come me e il senatore Caliendo, la critica che tutto questo nasce per sfiducia nei giudici. Non è così. mi rivolgo a chi muove questa critica - è che la sfiducia nei giudici, in particolare nell'esercizio del potere discrezionale sulla quantificazione della pena, afferiva esattamente alle due leggi che avevo richiamato, essendosi aumentati a dismisura i minimi della pena e quasi di poco i massimi, proprio perché si voleva, da parte del legislatore, non contento evidentemente dell'agire dei giudici, che le pene fossero tutte tali da poter aprire o spalancare le porte del carcere a chi quei reati aveva commesso e senza eccezioni di sorta. risponderà del reato di corruzione - com'è giusto che sia - che prevede al momento una pena di otto anni di reclusione. Quanto ciò sia ragionevole non è qui dato approfondire. Quindi, la critica - mi dispiace - non è esatta.

chi ha deciso di entrare in politica non può poi pretendere di rientrare in magistratura, conservando l'apparenza dell'imparzialità. In altri termini, riteniamo che avesse ragione Marx quando affermava - chiaramente edulcoro il termine - che non si può essere prostitute e vergini nello stesso identico tempo.

mi si deve spiegare il motivo per cui si prevede un reato specifico di corruzione in atti giudiziari, e cioè sostanzialmente un'ipotesi aggravata rispetto all'ipotesi normale di corruzione, e non si debba prevedere invece, ad esempio, l'ipotesi di una concussione commessa dal magistrato. Questo è possibile e a volte è anche accaduto, in specie, poi, se la corruzione in atti giudiziari ha un minimo e un massimo di pena assolutamente simili, e in un caso identici, al reato di concussione. Pertanto, non vi è chi non possa accorgersi che la identità di pena tra la corruzione in atti giudiziari e la concussione commessa da un magistrato prevede delle sanzioni tra di loro assolutamente contrarie alla ragionevolezza del sistema. Tutto qua, nient'altro che questo. Se esiste reato di corruzione in atti giudiziari, esiste perché si ritiene qualsiasi reato contro la pubblica amministrazione di gran lunga più grave di tutti gli altri, ove commesso con riferimento all'attività giurisdizionale.

vi è ragione alcuna per non chiudere il sistema e conseguentemente prevedere un'ipotesi aggravata per il reato di concussione e una serie di ipotesi aggravate

perché così si sarebbe data piena fiducia ai giudici che per ipotesi, attraverso il giudizio di equivalenza e prevalenza, possono agire sui meccanismi sanzionatori proprio attraverso questo giudizio. Certo, lo avremmo potuto fare, ma sarebbe stata una scelta in aperta contraddizione con l'ipotesi autonoma di reato che è la corruzione in atti giudiziari. Chi ha avuto modo di frequentare le aule di giustizia e di interessarsi di diritto, ovvero di interessarsi di diritto senza frequentare le aule di giustizia, ovvero di frequentare le aule di giustizia senza interessarsi di diritto, sa bene

non potevamo prevedere tutte queste ipotesi autonome di reato, e da lì necessariamente è scaturita la scelta di operare attraverso circostanze ad effetto speciale, e quindi circostanze tali da evitare, attraverso il giudizio di equivalenza o di prevalenza, un eccessivo abbassamento nella sanzione. Ma come potete immaginare che possano essere ugualmente gravi e non diversamente sanzionati i reati di corruzione, di millantato credito o di traffico di influenze che, invece che essere posti in essere da un cittadino qualunque, vengano commessi esattamente da quei soggetti che, per l'attività che svolgono (magistrati, avvocati, personale ausiliario dei giudici), hanno maggiore credibilità - penso in particolare al millantato credito o al traffico di influenze - o maggiore possibilità di accesso rispetto allo snodo decisionale? A me non sembra che tutto questo sia irragionevole e mi meraviglia - devo dire la verità - che, al di là evidentemente della la senatrice Lo Moro, che pure per un certo periodo di tempo

il secondo scopo di questa legge sia la tutela ad ogni costo della neutralità, anche in apparenza, dell'azione giudiziaria. Quando noi iniziamo a creare una serie di sbarramenti sanzionatori che riguardano determinati reati (corruzione, millantato credito e traffico di influenze) con riferimento all'azione del giudice, creiamo una deterrenza rispetto a quello che normalmente viene chiamato aggiustamento dei processi.

di quel fenomeno giudiziario riguardava per l'appunto le decisioni dei giudici. Sanzionare in maniera più più rilevantemente seria tutto ciò che in qualche modo possa toccare l'immagine del magistrato che deve decidere è un qualcosa a tutela del buon nome e del prestigio della magistratura. del buon nome e del prestigio della magistratura. Io non credo che possa essere seriamente tutelato il prestigio della magistratura se il

da chi ha la possibilità di avvicinare quel giudice per ragioni del tutto diverse dall'aggiustamento, e può farsi vedere dal cliente o dalla persona verso cui millanta in colloquio più o meno affabile con il giudice. Guardate che queste non sono cose che non esistono. Nel 1980 andai a fare una rogatoria in Francia e rimasi colpito dal fatto che i giudici non venivano assolutamente avvicinati da alcuno quando si muovevano nei corridoi o in prossimità delle aule di udienza. Ne chiesi la ragione e mi venne spiegato che o dovevano avere la scortesia di allontanare chi si avvicinava loro, ovvero non era opportuno quell'avvicinamento; il tutto a tutela dell'immagine, oltre che propria, della magistratura. Devo dire che io, in venticinque anni di carriera, non sono mai andato a prendere il caffè al bar, probabilmente perché avevo timore di tutto questo. Ma ritengo che chi afferma che quello in esame sia un provvedimento che si fonda sulla sfiducia dei giudici ovvero contro i giudici ha una lettura miope del testo e probabilmente non sa neanche da che parte stia di casa la tutela del prestigio della magistratura.

Onorevoli colleghi, la Presidenza, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, dichiara improponibili gli emendamenti 1.1, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 3.100, 3.0.100, 5.100, 5.0.100, 5.0.101 e 5.0.103, in quanto estranei all'oggetto del disegno di legge, che reca modifiche al codice penale esclusivamente con riferimento ai reati commessi nell'esercizio dell'attività giudiziaria. Passiamo all'esame degli articoli,

un Paese buono solo ad accogliere filibustieri di ogni provenienza. La corruzione, quindi, è un fenomeno che deve essere fortemente combattuto,

Il problema è che il fenomeno diventa più odioso se trova terreno fertile presso le aule di giustizia. Come correttamente ha detto il relatore, c'è l'aspettativa da parte dei cittadini

Questa aspettativa maggiore, che proviene da parte della cittadinanza quale aspettativa di civiltà, deve ovviamente comportare un aumento delle pene e una seria sanzione nel caso in cui gli operatori del mondo della giustizia si distacchino dal principio della legalità. Forse è un atteggiamento quasi utopistico, ma chi opera nel mondo del diritto sa che le procedure si chiamano riti, riti, quasi a voler richiamare una funzione che ha implicazioni quasi religiose. Forse il tribunale deve diventare un luogo sacro, e così deve essere. essere. Nel momento in cui sorge il dubbio sull'operato della magistratura, sull'operato del tribunale e di chi lavora nella giustizia, signori, crolla l'impianto della giustizia.

È una di quelle ombre che possono destituire l'impianto di una civiltà e di una cultura giuridica. Quindi, l'indipendenza della magistratura non deve essere solo rispetto ai poteri legittimi. Deve essere soprattutto un'indipendenza e un distacco da quelli che sono i poteri illegittimi e sicuramente dal fenomeno corruttivo. Per questo ben venga il disegno di legge

su quasi tutti i provvedimenti sulla giustizia approvati, in particolare, in quest'ultima legislatura.

non c'è una risposta repressiva e viene poi meno anche l'efficacia dissuasiva della norma. Per questo è inutile prevedere aggravamenti di pena e circostanze aggravanti se poi

agli arresti e alle immediate liberazioni, a chi non va in galera, a chi effettivamente non subisce la pena che gli spetta*. (Applausi *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, signori senatori, ci troviamo ad affrontare questo disegno di legge e devo dire che, con tutti i problemi che ha il pianeta giustizia, mi verrebbe proprio da ridere, non da sorridere. Con tutti i temi che abbiamo ancora all'esame della Commissione giustizia e dell'Assemblea e che hanno a che fare con il settore (corruzione, prescrizione, lotta alla criminalità, codice antimafia, processo civile, giudici di pace, giudici onorari)

si riesce a capire che c'è una deviazione di attenzione verso i controllori e che si cerca di scaricare responsabilità che sono di altri (della politica ma non solo) su coloro che dovrebbero semplicemente applicare la legge,

Non vorrei che venisse data un'importanza capitale a questa modalità di trattare il tema della giustizia. Infatti, dal punto di vista del diritto sostanziale e del diritto penale, ancora una volta si pensa di poter risolvere i problemi della giustizia soltanto con l'aumento delle pene. Invece di far funzionare gli uffici giudiziari, gli uffici delle procure, gli uffici dei giudici, le segreterie, le cancellerie, di fare in modo che il Consiglio superiore della magistratura stesso sia in grado di intervenire e di verificare cosa fanno i giudici, invece di adottare gli strumenti che consentano una verifica, anche preventiva, dell'attività non solo giurisdizionale, ma anche giudiziaria, si pensa di risolvere il problema della

corruzione, concussione - a mio modo di vedere bisogna condannarlo a dieci volte la pena, non aumentargliela della metà. È grave dal punto di vista istituzionale che si possa verificare un fatto del genere, però è ridicolo che si intervenga in questa maniera. Facciamo funzionare i sistemi di controllo all'interno della magistratura, facciamo funzionare i meccanismi del Consiglio superiore della magistratura e soprattutto facciamo in modo che venga data la possibilità di lavorare. Concludo questo mio breve intervento - perché credo che questo disegno di legge non meriti molto più tempo - ricordando a tutti noi, a me stesso per primo: trattiamo i veri temi della giustizia, quelli legati alla criminalità organizzata, al codice antimafia (che ancora nelle secche della Commissione giustizia e speriamo che venga al più presto in Aula), al processo civile, alla riforma dei giudici onorari e dei giudici di pace e a tutti gli altri temi che sono bloccati all'interno della Commissione giustizia. In questo modo faremo certamente qualcosa di utile per il Paese e anche qualcosa di onorabile per questo Parlamento. in sede di discussione generale, ho concentrato la mia attenzione sulla figura professionale del giudice e quindi su uno dei destinatari del provvedimento,

di un ordine degli avvocati e l'ho trattenuta per circa dieci anni, accolgo con molto favore il provvedimento in esame, perché la figura dell'avvocato aveva nel passato e ha avuto sempre nella storia una

promotore di un pensiero filosofico nel nostro Paese. Essere avvocato è qualcosa di importante. Quando si prevede, come fa il

per ridare autorevolezza e per costituire e rappresentare una sorta di deterrenza alla commissione di certi reati, che sono odiosi, innanzitutto perché con il millantato credito si getta un'ombra anche sulla figura del giudice. Sono dell'avviso che il giudice non possa essere ombrato da alcunché. Il giudice, prima di essere

certamente il provvedimento in esame non introduce un cambiamento epocale nel nostro codice penale ed è evidente che non è contro i magistrati.

che anche coloro che sono chiamati a giudicare i cittadini e quindi si pongono in una posizione più alta possono commettere reati gravi, come la corruzione e la concussione.

contrariamente ad altri provvedimenti di minor importanza, che hanno impegnato per giorni la nostra Assemblea, esprimo il convinto voto favorevole del Gruppo per le Autonomie-Partito socialista-MAIE, perché

Signor Presidente, sarò davvero brevissimo nell'intervento in cui dichiaro l'adesione del mio Gruppo al provvedimento, che si pone in sintonia e in grande coerenza con altri interventi di vasto raggio in tema di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione: la corruzione, la concussione e tutto l'insieme di questi reati. Si pone in coerenza proprio perché rende più severa la deterrenza nei riguardi degli odiosi reati di questa natura contro la giustizia e contro

dedicato alla funzione importantissima ed essenziale di applicare la legge con equità e giustizia. Mi sento di poter dire che questa norma, che apparentemente sembra essere, come è stato sollevato da che induce elementi di sfiducia nei riguardi della categoria togata (sia essa di magistrati, di operatori del diritto o di difensori e patrocinanti quali sono gli avvocati), è invece posta a tutela della loro dignità perché li protegge dalle insidie che possono esservi in situazioni molto complesse, quali quella del giudicare, e dalle influenze che possono essere esercitate - a volte accade perniciosamente - proprio su chi ha anche la piena autonomia e l'assoluta discrezionalità - in molti casi esente da interventi disciplinari - nell'applicare e interpretare le norme e nel valutare le prove. Del resto, già in discussione generale, con qualche notazione critica, si è visto che nell'approvazione dei singoli articoli vi è stata una larghissima maggioranza.

Giovenale: «*Quis custodiet ipsos custodes?».* Noi rispondiamo: è per dare tutela a chi è custode della legge che gli diamo gli strumenti perché possa meglio esercitare la sua funzione.

In questo caso si aggiungono altre aggravanti per quanto riguarda la concussione e anche per quanto riguarda altre ipotesi riguardanti il favorire o il danneggiare una parte in processo o il delitto di il delitto di traffico d'influenze illecite, ma stiamo parlando, appunto, di aggravanti che si innestano su un meccanismo di notevole aumento delle pene. possiamo dirci soddisfatti del fatto che affrontiamo un fenomeno così grave, che colpisce la nostra società, come quello della corruzione, solo e unicamente con l'aumento delle pene? Io penso di no;

amministrare la giustizia in modo assolutamente imparziale ed essere una garanzia per i cittadini, è certamente un fatto, dal punto di vista sociale, politico e proprio della fiducia dei cittadini

Detto ciò, non vorrei però che questo provvedimento fosse accompagnato da un'enfasi e anche da una interpretazione politica.

che questo provvedimento possa essere interpretato da qualcuno come una sorta di vendetta nei confronti della magistratura, quasi una contrapposizione

diventare una bandiera o uno strumento di aggressione nei confronti di un altro potere dello Stato. Ahimè ci dispiace - nel riconfermare nel riconfermare le valutazioni che abbiamo fatto all'inizio - che questo disegno di legge arrivi a un aumento notevole delle pene, assolutamente in scia purtroppo con la tendenza che c'è stata

Qualcuno ha citato l'omicidio stradale, ma potrei citare molti altri

da parte di chi si trova in quegli uffici e in quelle stanze dove si amministra la giustizia e dove la corruzione deve essere combattuta: ciò tradisce un impegno morale, giuridico e civile e deve essere sanzionato severamente, in maniera anche più severa rispetto al normale cittadino. Non possiamo che convenire su questo, proprio noi forza politica che alla legalità facciamo un richiamo continuo e

fatto che la lotta effettiva alla corruzione va fatta non solo con questi provvedimenti che oggi stiamo votando e che incidono in maniera del tutto residuale nell'ambito del fenomeno complessivo, ma anche dando alle forze investigative e alla magistratura

macchina della giustizia, ma anche il fatto obiettivo che certe condotte vengono scoperte a distanza di anni dai fatti. Anche se la prescrizione non operasse in assoluto, noi non saremmo contenti se una sentenza di condanna, e tanto più una di assoluzione, arrivassero a distanza di

Tornando a quello che stavo dicendo, non possiamo non convenire sul disvalore sociale dei reati di concussione, induzione indebita, millantato credito e traffico di influenze illecite, e non possiamo che convenire che la sanzione debba essere maggiormente se commessa da certe categorie di persone. Così come, nel caso della corruzione per atti giudiziari, che già punisce il pubblico ufficiale che favorisce una parte processuale, riteniamo che debba essere responsabile anche il corruttore e debba essere sanzionato più gravemente qualora quel corruttore, cioè la parte attiva

previsto anche da una Convenzione dell'ONU del 2000 che l'Italia ha sottoscritto e che invita gli Stati membri a porre in essere operazioni sotto copertura anche per combattere il fenomeno corruttivo), l'estensione del cosiddetto Daspo per i politici (l'interdizione e l'incandidabilità

Infine mi piace fare un richiamo, perché ho avuto l'impressione che fosse una sorte di *karma* che torna in quest'Aula a distanza di decenni: il senatore Palma prima ha invitato tutti noi a fare un salto indietro nel passato di vent'anni ed effettivamente, facendo questo salto temporale in tema di corruzione in atti giudiziari, viene alla mente proprio la nota vicenda che ha visto il giudice Metta

con riferimento a Mondadori. Quindi, quasi per un sorta di *karma* cosmico, adesso non possiamo che essere soddisfatti che questa iniziativa legislativa porti la prima firma proprio di un esponente di quel partito

malati con quella parte della magistratura, che non va idealizzata in toni eroici - perché sappiamo che il buono e il cattivo c'è in ogni settore sociale - ma va messa nelle condizioni di operare correttamente e svolgere bene il suo lavoro.

devo dire che il provincialismo imperante del dibattito nel nostro Paese si è rivelato anche oggi, focalizzata l'attenzione come se questo provvedimento avesse l'obiettivo di colpire l'eventuale magistrato che commettesse questi reati. Forse non avete la consapevolezza che, grazie a Dio, nel nostro Paese non c'è un numero apprezzabile di magistrati che abbia commesso reati di questo tipo;

e quindi do ragione alla senatrice De Petris quando critica il Parlamento quando aumenta le pene, perché sono molto più favorevole e convinto dell'utilità della certezza della pena.

qualcuno che invece dovrebbe esserne immune per la sua scelta di vita e per il giuramento che ha fatto all'inizio della professione. Se leggete

non è un provvedimento che vuole colpire un determinato episodio, ma vuol dare all'architrave del nostro sistema penale un'immagine di coerenza, di parità dei diritti, di parità delle responsabilità, di parità nella valutazione dei comportamenti. Quando c'è una diversità, a quella diversità corrisponde una diversa valutazione. Questa è la logica di questo provvedimento,

che non esistono - o, se esistono, sono uno su 10.000 - reati di questo tipo commessi da magistrati o da appartenenti all'amministrazione giudiziaria.

provvedimento sia arrivato in Aula, perché quantomeno diamo quella possibilità di lettura del nostro sistema penale tale da garantire i principi fondamentali della Costituzione.

dare una risistemazione al sistema penale, che è stato squilibrato con determinate pene. Ecco perché occorre questo provvedimento. Concludo. Credo che la votazione dei vari articoli all'unanimità stia a significare una sola cosa:

Era necessario se questa possibilità, questa idea, questa posizione del magistrato e dell'operatore giudiziario in genere veniva ad essere dimenticata e quindi ciò poteva essere oggetto di eventuale critica. Basta questo perché una norma sia necessaria, perché quando si ravvisa la non completezza della norma norma e che il sistema consente una falla, vuol dire che vi è necessità di un intervento, ed è questa la ragione per cui voteremo a favore di questo provvedimento. Signor Presidente, colleghi, la lotta alla corruzione deve impegnare il Paese, e con esso il Parlamento, con rigore, serietà ed equilibrio.

va sviluppata con una dimensione progettuale che deve contenere un vero e proprio approccio integrato repressivo-giudiziario - sì, senz'altro - e da questo punto di vista il Parlamento, in questa legislatura, ha fatto dei passi in avanti. L'aspetto preventivo è anch'esso una dimensione dell'approccio integrato che non va assolutamente sottovalutate; una dimensione che è cresciuta con l'Agenzia anticorruzione. Finalmente nel nostro Paese questa dimensione si sta scoprendo, ma ha bisogno anch'essa di fare notevoli passi in avanti. Non possono mancare, in un approccio integrato, i comportamenti sociali e culturali; deve diventare convinzione dei cittadini che la corruzione non è una scorciatoia, ma una rovina, un danno per se stessi e per il Paese. approccio integrato non può trovare nel Parlamento divisioni strumentali e non può trovare nella politica ritardi o strumentalizzazioni. questo provvedimento non va sopravvalutato e non deve diventare l'occasione per degli scontri o per delle rivincite nella società nei confronti dei soggetti impegnati nel campo giudiziario (il Partito Democratico non si presta a questo uso); tantomeno esso deve essere sottovalutato o svilito. È un provvedimento che prova a coprire un tassello che mancava nella maggiore organicità che abbiamo iniziato a produrre nel campo della lotta ai reati che fanno parte del novero della corruzione e che riguarda l'esercizio delle attività giudiziarie. Se scorrete i pochi articoli, che lo troverete il continuo riferimento all'esercizio delle attività giudiziarie che comprende tutti i soggetti che fanno parte di tali attività: i attività: i magistrati, gli avvocati, gli ausiliari del giudice, ma anche tutto il personale amministrativo degli uffici giudiziari, com'è stato ben chiarito con un emendamento del relatore che pochi minuti fa abbiamo approvato all'unanimità. Ecco perché non si può astrarre un soggetto e pensare che questo provvedimento possa essere punitivo, ad esempio, nei confronti dei magistrati. L'esercizio dell'attività giudiziaria è delicatissimo

Signor Presidente, voglio portare all'attenzione di quest'Assemblea l'ennesima vertenza del mondo del lavoro. Parlo del salumificio Spiezia di San Vitaliano di Nola parlo, naturalmente, dei suoi lavoratori e delle loro famiglie che da tre mesi non percepiscono stipendio e, nonostante tutto, stanno lottando con tutte le forze per difendere il loro posto di lavoro messo in pericolo per la chiusura dell'azienda. Presidente, parlo di 90 lavoratori, 90 persone in carne ed ossa, con un'età media di cinquant'anni, con mogli e figli a carico, per non parlare dei mutui da pagare. Parlo di scongiurare l'ennesimo disastro sociale nel Sud. Ho ascoltato le voci dei lavoratori in un video nel quale sono state avanzate proposte intelligenti e fattibili che saranno portate venerdì prossimo all'incontro al MISE. chiedono alla politica di non essere abbandonati ed essere aiutati a non far morire la loro fabbrica che, se aiutata, si potrebbe salvare ed essi potrebbero quindi continuare

positive in merito, perché hanno fatto delle proposte veramente intelligenti che possono salvaguardare 90 posti di lavoro, nell'interesse loro e delle rispettive famiglie. Spero veramente che le loro richieste vengano accolte.

In Sicilia il posto di lavoro è qualcosa non facile né da acquistare, né da acquisire, né da riacquisire una volta perduto.

di maggioranza relativa - di lasciare che le cose vadano così come devono andare, con i più forti che impongono la propria volontà e i più deboli che accettato la volontà

Se la politica decide di chiudersi in un camerino, poi non può lamentarsi di non poter correre i 100 metri. Se ci diamo come regola quella di lasciare che il mercato del lavoro si autoregoli e di sottrarci a un condizionamento che è dovuto per Costituzione, a questo punto la responsabilità politica è piena e ricade su di noi. Essa è piena soprattutto nei confronti di quella parte di questo emiciclo che si definisce di sinistra - non ho capito a che titolo - e lascia che ciò avvenga. avvenga. Capisco quei lavoratori che hanno accettato di vedersi ridurre gli emolumenti che avevano già maturato. Ripeto, lo capisco. Non capisco invece il silenzio delle forze politiche che dovrebbero evitare che queste cose accadano. Signor Presidente, colleghi, vorrei oggi richiamare la vostra attenzione sulla difficile condizione che da tempo caratterizza la quasi totalità degli 8.000 dirigenti scolastici italiani, che hanno visto le responsabilità connesse al loro ruolo aumentare esponenzialmente. Emblematico è quanto accaduto alla preside Franca Principe dell'Istituto «Carlo Pisacane» di Sapri, presso il quale svolge il proprio compito da nove anni, migliorandone nel tempo la struttura (in origine decisamente compromessa), la forma organizzativa, la qualità del servizio, interpretando i bisogni di un territorio di certo non facile e assumendosi la responsabilità collettiva di circa 900 studenti e di oltre 100 dipendenti. luglio 2011 alcuni studenti dell'istituto, intenti a sostenere l'esame di maturità, sono riusciti ad accedere a un lastrico solare, normalmente inaccessibile e non destinato ad altre attività se non quelle di manutenzione, lasciato aperto e incustodito da una collaboratrice scolastica dell'istituto, nonostante fosse stato espressamente richiesto dalla dirigente di rendere inaccessibile quella zona. In questa circostanza uno degli studenti è precipitato dal lastrico, riportando lesioni dalle quali, fortunatamente, si è completamente ripreso. Nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria la collaboratrice scolastica responsabile della negligenza, che ha ottenuto il prepensionamento, non è stata indagata perché dichiarata inidonea al servizio, mentre l'ente proprietario, tenuto alla manutenzione, è stato assolto. L'unica a pagare per quanto accaduto è stata la preside, oltretutto assente quello sfortunato giorno in quanto impegnata a presiedere una commissione di esame presso un altro istituto, che è stata condannata a un mese di carcere e a un risarcimento di 15.000 euro a titolo di provvisionale provvisoriamente esecutiva. Colgo quindi questa occasione per ricordare che la responsabilità oggettiva connessa al ruolo non può *tout court* essere trasformata in colpa, dolo e che, pertanto, il decreto legislativo n. 81 del 2008 deve essere assolutamente modificato. Non è ammissibile che i dirigenti scolastici paghino per responsabilità di inadempienze di altri enti o di altri soggetti professionali. Concludo esprimendo tutta la mia solidarietà a Franca Principe e a questa categoria professionale che giustamente protesterà domani manifestando qui a Roma.

di quattro operai impiegati, fino a metà settembre 2016, presso la Fincantieri SpA di Monfalcone e licenziati a causa di una sospensione lavorativa al di fuori della pausa consentita nella notte tra il 14 e il 15 settembre 2016. Dopo il licenziamento, i quattro lavoratori si sono rivolti al giudice del lavoro che, costatando che non vi era recidiva a loro carico, poiché non sussistevano indicazioni scritte sulla collocazione della pausa di lavoro in una determinata fascia oraria, e che la stessa Fincantieri aveva ammesso che una flessibilità nell'orario di pausa era possibile, aveva ordinato l'immediato reintegro dei lavoratori, in piena applicazione dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori nella più recente versione. Sta di fatto che ad oggi questo non è ancora

per se stessi e per gli altri e ha deciso di non dare seguito al reintegro fisico sul posto di lavoro dei quattro operai, interdicendo loro l'attività lavorativa, limitandosi al reintegro formale nell'organico e alla corresponsione - quella sì - dello stipendio, degli arretrati, delle previdenze e assicurazioni pregresse.